Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, con il provvedimento in esame il Senato è chiamato ad autorizzare la ratifica e l'esecuzione di una serie di accordi internazionali in materia ambientale, fatti tra il 1991 ed il 2015. Essi, da un lato, pongono a carico del nostro Paese alcuni obblighi, soprattutto per le considerazioni ambientali e sanitarie da includere nella preparazione dei piani e programmi in un contesto transfrontaliero, ma, dall'altro, aprono la via ad una maggiore cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, con particolare riferimento alla lotta all'inquinamento nel Mediterraneo, mare praticamente chiuso e ad alta densità di navigazione, nel quale quindi gli incidenti sono più probabili e potenzialmente più difficili da gestire. La ratifica dell'emendamento di Doha è un atto dovuto per proseguire gli impegni presi dall'Unione europea per il secondo periodo del Protocollo di Kyoto, per gli anni 2013-2020, attraverso un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas serra. L'emendamento di Doha non comporta nuovi impegni per il nostro Paese né per tutta l'Unione europea rispetto a quelli fissati nel pacchetto sul clima, cosiddetto Pacchetto clima-energia, finalizzato a raggiungere entro il 2020 i cosiddetti obiettivi 20-20-20, cioè riduzione delle emissioni di gas sera, aumento dell'energia da fonti rinnovabili e miglioramento dell'efficienza energetica. Purtroppo, il secondo periodo di impegni (2013-2020) riguarda solo il 14 per cento delle emissioni globali, dal momento che soltanto gli Stati membri dell'Unione, altri Paesi europei e l'Australia si sono impegnati in tal senso, mentre gli Stati Uniti, la Russia, il Canada, il Giappone e i Paesi in via di sviluppo non hanno assunto impegni. Secondo gli scienziati che lavorano con l'ONU, una riduzione così modesta spingerebbe le temperature addirittura ad un aumento di tre gradi, proprio all'opposto degli obiettivi che occorre raggiungere per contenere i cambiamenti climatici. In questo periodo le nostre imprese sono state impegnate ad adottare accorgimenti tecnologici dispendiosi per abbassare le emissioni di CO2, senza risultati concreti, vista la poca rilevanza dell'ammontare delle emissioni risparmiate a livello mondiale. Il nostro voto, che nel complesso sarà favorevole al provvedimento, si riferisce soprattutto alla prospettiva di fiducia per il nuovo accordo sul clima raggiunto recentemente alla XXI Conferenza delle parti a Parigi, applicabile a tutti i Paesi per il periodo successivo al 2020. Per la prima volta si è raggiunta un'adesione vincolante anche da parte di Stati che in passato si sono dimostrati contrari agli accordi internazionali con l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei due gradi rispetto ai livelli precedenti alla rivoluzione industriale. Sappiamo adesso che avremo una Strategia nazionale, in accordo agli obiettivi mondiali, per uno sviluppo a basse emissioni di carbonio; è un fatto in sé positivo, ma che poco dice rispetto alla strada che verrà intrapresa per tradurlo in fatti concreti:

Coloro che governeranno potranno metterci di tutto, circostanza che forse alcuni giudicheranno preoccupante, ma che a noi pare invece garantire la flessibilità che occorrerà al momento giusto per rivedere alcuni aspetti della politica energetica, quando torneremo ad amministrare il Paese.

in materia ambientale legati all'attuazione del Protocollo di Kyoto. All'ISPRA spetterà altresì il compito di raccogliere i dati ed aggiornare il sistema utilizzato per archiviarli. Naturalmente,

non abbiamo motivi particolari per opporci alla ratifica di questi sei accordi in materia ambientale. Auspichiamo soltanto che il rispetto dei limiti imposti da questi accordi sia sia effettivo da parte di tutti gli Stati firmatari, perché la salvaguardia e la tutela dell'ambiente e dei cosiddetti beni globali comuni non può essere l'affare di pochi: deve essere un dovere di tutti. Gli oneri non sono

che preveda, con obiettivi scadenzati, la neutralità emissiva e la decarbonizzazione. Ora però questo è il punto: qui ci sono stati tutti voti a favore, ma le politiche di questo Governo sono ben lontane dal perseguire questa strada. Quindi, è bene che anche in sede di dichiarazione di voto si squarci questo velo di ipocrisia, perché domenica prossima andremo a votare per un *referendum* e questo Governo, che

provocato dalle navi e di lotta all'inquinamento del Mediterraneo. È vero che il testo è concentrato soprattutto sulla prevenzione dell'inquinamento da navi, ma, anche in questo caso, è impossibile non far riferimento alla questione delle trivellazioni. Lo dico in modo molto chiaro: i dati dell'ISPRA pubblicati nel 2014 dicono che nel nostro mare ci sono 200.000 imbarcazioni di grandi dimensioni, tra traghetti, cargo e imbarcazioni commerciali, di cui circa 300 navi cisterna che giornalmente trasportano prodotti petroliferi. quindi il Mediterraneo subisce sversamenti di idrocarburi per circa 600.000 tonnellate e sono da registrare 27 incidenti occorsi nel Mediterraneo. Quel Protocollo aspettava di

viene anche sottolineato che ci sono 125 milioni di tonnellate di idrocarburi, circa il 10 per cento degli idrocarburi mondiali, che vengono movimentati ogni anno nei porti italiani. doppiamente allarmante il fatto che si voglia lasciare alle imprese petrolifere la possibilità di continuare ad estrarre idrocarburi liberamente nel nostro mare, dilatando a non finire i tempi per il *decommissioning* delle piattaforme. sul tema delle piattaforme abbiamo presentato un'interrogazione sulla base di dati molto allarmanti arrivati da una ricerca del WWF. casi di sversamento e molte questioni aperte. Dico questo per dire che è molto labile l'idea che si possa affermare, anche votando a favore, che il Governo si stia impegnando per la lotta all'inquinamento del mare, perché quanto sta accadendo in questi giorni quello che è emerso dalle inchieste ci dicono esattamente il contrario. La stessa questione riguarda il tema delle consultazioni pubbliche e la partecipazione dei cittadini alle questioni ambientali, che viene trattato dalle norme relative alla Convenzione di Espoo tra la Commissione economica europea e le Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale

e alcuni sono già superati da altri accordi che dovremo andare a ratificare a breve. Questo, come veniva detto da altri colleghi, è il sintomo della poca attenzione del nostro Paese: laddove molto spesso alle parole non seguono i fatti, agli accordi non seguono le ratifiche. Inoltre, questi accordi, dopo aver giaciuto per anni, vengono accorpati e costretti in un'anomala procedura che umilia, ancora una volta, il dibattito parlamentare, perché abbiamo la fretta di dover ratificare in vista all'accordo di Parigi, da firmare a brevissimo a New York. Ci troviamo, quindi, di fronte alla ratifica di accordi superati nei numeri e nei fatti. Sono Sono contenta che il Governo abbia voluto accettare gli ordini del giorno su due dei temi che riteniamo più importanti, di cui alla lettera *a)* e alla lettera ma quanti ordini del giorno sono stati accolti da questo Governo senza che poi ne sia stato dato alcun seguito? Questo ci preoccupa e per questo ci importa andare ancora a sottolineare l'importanza di questi ordini del giorno. L'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, di il Protocollo di Kyoto è l'unico trattato internazionale in vigore finalizzato a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e quindi costituisce un impegno fondamentale ed importantissimo. ed importantissimo. Proprio al fine di assicurare la continuità dell'azione di quel primo Accordo, che copriva il periodo 2008-2012, si è andati a firmare un secondo Accordo, l'emendamento

Sebbene, come evidenziato, il Pacchetto clima-energia abbia già superato questi dati, non siamo neanche andati a verificare nelle opportune sedi se gli obbiettivi del Protocollo di Kyoto e dell'emendamento di Doha quali siano effettivamente i risultati di tali accordi. È quindi assolutamente necessario attuare queste verifiche e renderci conto che questo è un punto di partenza e non può essere un punto di arrivo.

anche per l'Italia e per gli altri Paesi che non lo hanno ratificato, nel marzo del 2004, quando sei Paesi dell'Unione lo hanno ratificato. Il Protocollo prevedeva obblighi vincolanti anche per quanto riguarda l'adeguamento legislativo e normativo dei Paesi, ma noi non abbiamo fatto nulla, abbiamo preso degli impegni a cui non abbiamo

che sappiamo ammontare al dieci per cento del totale. Quindi, come vogliamo salvaguardare il nostro mare, quando sono quattordici anni che non ci siamo occupati di ratificare questo importante Patto di La Valletta?

il ricorso ad un solo strumento legislativo attraverso cui si procede alla ratifica e all'esecuzione cumulativa di più atti di grande importanza, i quali richiederebbero ciascuno un proprio specifico provvedimento di ratifica. Riteniamo altresì operativamente inadeguato l'inserimento del Capo II, che introduce le norme di adeguamento all'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto e non perché nutriamo particolari riserve in merito alla necessità di procedere con atti concreti di programmazione. Proprio ieri infatti, in sede di discussione delle mozioni sull'ecobonus, ho evidenziato l'assenza di un'adeguata programmazione di settore, specifica, coordinata, approfondita e trasparente. Ne avremmo, però, preferito una trattazione separata, nell'ambito di un apposito disegno di legge non frettoloso, il cui *iter* non fosse obbligato al rispetto di tempi strettissimi cui ci costringe il Governo, svilendo il ruolo delle Camere ed esautorando, giorno dopo giorno, le prerogative che la Costituzione vigente attribuisce alle Aule parlamentari. Anche questa volta, nulla accade per caso: probabilmente siamo di fronte a un'accelerazione imposta affinché il Governo possa recarsi a New York il prossimo 22 aprile per sottoscrivere l'Accordo di Parigi sul clima. La mancata ratifica dell'emendamento di Doha potrebbe costituire, infatti, un impedimento per la regolare sottoscrizione da parte del Governo italiano dell'accordo predisposto nell'ambito di COP 21. D'altra parte, gli accordi che l'Assemblea è chiamata a ratificare sono importanti e devono essere inseriti nella filiera delle azioni che il nostro Paese è tenuto ad adottare nel campo energetico, nel contrasto ai cambiamenti climatici e nelle procedure di VIA, in particolare andando a predisporre la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni, all'interno della quale definire indirizzi e azioni utili per la trasformazione della società italiana, l'innovazione tecnologica e l'efficienza in vari settori, individuando, inoltre, compiti e limiti operativi dei soggetti chiamati all'attuazione. Pertanto, con il consueto senso di responsabilità che contraddistingue l'operato del nostro Gruppo, sosteniamo con favore l'adozione del provvedimento in esame, ancora puntualizzando il disagio nel proseguire il nostro operato all'interno di una cornice così frammentata e priva di un chiaro quadro generale di riferimento, alla definizione del quale auspichiamo possano partecipare attivamente, nel prossimo futuro, tutti i senatori e le Commissioni interessate, senza limiti di tempo. Dichiaro, perciò, il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

evidenziare che i nostri ritardi, che spesso sono più politici che non di fatto, non corrispondono al Paese che in molti interventi ho sentito descritto: siamo un Paese più in regola di molti altri Paesi europei e di molti Paesi industrializzati, sia in termini di emissioni, sia in termini di rispetto degli obiettivi che ci siamo dati con il Protocollo di Kyoto. Siamo un Paese che percorre regolarmente la propria strada verso le energie rinnovabili più di quanto abbiano fatto altri Paesi. Allora, con minore senso di colpa

aggiungo che abbiamo fatto bene a votare in modo separato sull'articolo 1, come ci è stato consigliato, perché si tratta di argomenti differenti, contenuti in un unico articolo, che dovevano essere analizzati separatamente, così come il senatore D'Alì ci ha indotto a fare, credo, giustamente.

una mancanza di risposte in percentuali adeguate al numero di interpellanze, interrogazioni e mozioni che sono state presentate.

attraverso il quale possono conferire con il Governo, e si esercita attraverso: "interrogazioni", per ricevere informazioni o chiarimenti su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo; "interpellanze", che chiedono conto nella domanda rivolta al Governo dei motivi o degli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale;». Era doveroso specificare di cosa parliamo. «Per ognuno degli strumenti vi è una tempistica da rispettare, ai sensi del Regolamento del Senato, al fine di fornire risposte ai parlamentari che le richiedano, che va da un massimo di 15 giorni, per le interrogazioni a riposta orale, ad un minino di un giorno per le interrogazioni con carattere d'urgenza, e da un massimo di un mese, per le interpellanze, ad un minimo di 15 giorni, per le interpellanze con procedimento abbreviato; il Regolamento, al Capo XIX, articoli da 145 a 161, dispone quanto sopra e altresì che, per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale e delle interpellanze, sia destinata, di norma, almeno una seduta per ogni settimana; ad oggi, la percentuale degli atti che hanno ricevuto risposta è di circa il 19 per cento» - al massimo, da altre indagini che ho fatto, si arriva al 22-23 per cento - «con un tempo medio di 126 giorni». La classifica dei destinatari vede all'apice il Ministero dell'interno con 820 atti ricevuti, quindi la Presidenza del Consiglio dei ministri

comunque molti Ministeri vengono coinvolti da interrogazioni e interpellanze. «Per molti parlamentari l'atto di sindacato ispettivo è l'unico strumento attraverso il quale interagire con il Governo e, ad oggi, molti di questi rimangono privi di risposte su questioni di carattere territoriale, che trattano tematiche sensibili per la cittadinanza; nel rispetto della centralità del Parlamento, i riformatori dei Regolamenti parlamentari, nel 1971, intesero rafforzare notevolmente» - e non a caso - «l'esercizio dell'attività di controllo parlamentare nei confronti del Governo. Pertanto, la situazione esposta è inaudita e inaccettabile, perché, di fatto, priva i parlamentari della funzione di controllo attribuita loro dalla Carta costituzionale. Considerato che: il primo firmatario del presente atto di indirizzo» ovvero il sottoscritto «si è avvalso dello strumento dell'interpellanza con procedimento abbreviato, disciplinata dall'articolo 156-*bis* del Regolamento del Senato, presentando in data 5 marzo 2015 l'atto di sindacato ispettivo 2-00252, con il quale denunciava la mancata risposta ad interrogazioni ed interpellanze da parte del Governo; detta interpellanza con procedimento abbreviato è stata sottoscritta da senatori

a dimostrazione del fatto che è diffusa l'insoddisfazione nei confronti del Governo; a distanza di oltre 5 mesi, non è stata fornita alcuna risposta da parte dell'Esecutivo e a tal proposito il primo firmatario

al punto tale da correre il rischio di diventare quasi ridicolo, perché l'azione era volutamente e ripetutamente rimarcata. «Nonostante i «Nonostante i molteplici interventi, in Aula non vi è stata, da parte del Governo, né alcuna risposta agli atti di sindacato ispettivo né alcuna presa di posizione in merito alla perdurante e annosa questione del basso indice di risposta agli stessi; basso indice di risposta agli stessi; senza il predetto strumento, il potere legislativo è, di fatto, privato della propria prerogativa di controllo sull'operato dell'Esecutivo e, quindi, vi è una forte divergenza tra quanto disposto dalla Costituzione e quanto in effetti realmente si verifica; sussiste quindi l'improcrastinabile necessità e urgenza che il Governo si renda pienamente consapevole del precedente che si sta consolidando,

possano smaltire l'arretrato di atti di sindacato ispettivo, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e della funzione di controllo riconosciuta ai parlamentari, dando conto, anche sinteticamente, di eventuali mancate risposte.

ma nel contempo, se esprimo questa soddisfazione e, se vogliamo, anche emozione, esprimo anche molta preoccupazione, perché mai riuscirei a perdonarmi e a perdonare al Governo, qualora questa mozione venisse accettata, se si perdurasse con il vecchio sistema. A quel punto, signor Presidente e onorevoli colleghi, chiederei con un tono se vogliamo un po' ironico ma non più di tanto, di cambiare il Regolamento di questo Senato e aggiungere un articolo che coincide con un noto aforisma:

Signor Presidente, ringrazio il senatore Amidei per la sua brillante e appassionata illustrazione. Io aggiungerò alcuni elementi a quanto affermato dal collega

e predisponemmo un'interrogazione parlamentare per chiedere perché il Governo non rispondeva alle interrogazioni parlamentari. Ebbene, il risultato è stato paradossalmente che a quell'interrogazione parlamentare ovviamente non abbiamo avuto risposta: qui sta il paradosso dal quale prende avvio questo momento.

Spesso siamo incappati in risposte, anche da parte di enti e amministrazioni,

L'unico dato importante che vorrei sottolineare è la sperequazione presente nelle percentuali di risposta: al Senato abbiamo un totale di risposte agli atti di sindacato intorno al 23,5 per per quanto riguarda gli atti presentati alla Camera siamo intorno al 37,3 per cento. E ciò mi fa venire in mente un'altra cosa. Questo dovrebbe essere un elemento aggiuntivo

sono riconducibili a una scarsa attività del Governo, che ha risposto in una certa percentuale, perché potrebbe ribattere che, effettivamente, il numero e la mole degli atti presentati sono

ciò che ritiene più utile. Ma è anche vero che non esiste alcun tipo di controllo da parte dei Gruppi parlamentari. E questo si ricollega a un altro discorso che ho già fatto in quest'Aula.

ai deputati e ai senatori viene lasciata la libertà di poter presentare qualsiasi tipo di atto, per cui si va da famigerati atti di sindacato ispettivo - famosi quelli

(si vede un comunicato stampa e si presenta subito un'interrogazione parlamentare, magari solo per apparire sui giornali per qualche minuto). Questa è sicuramente una prassi negativa che ogni Gruppo parlamentare avrebbe

un argomento basilare della vita democratica di un Paese. Stiamo parlando dei rapporti tra Parlamento e Governo. Il Parlamento è l'espressione della sovranità popolare, gestito per mandato elettorale. La vita democratica di uno Stato di diritto e di un Paese democratico si basa esclusivamente sulla centralità del Parlamento. Il Governo è un prodotto - non un sottoprodotto, ma un prodotto - del Parlamento, e infatti deve rimanere in carica e poter godere della fiducia

Il Governo ha residuali poteri legislativi in Costituzione. Solo in casi di necessità e urgenza, il Governo può sostituirsi al Parlamento, il quale Parlamento deve poi ratificare tutto il lavoro: o convertire quegli atti o modificarli o bocciarli. Qui, invece, siamo chiamati sempre più impellentemente a discutere di provvedimenti del Governo,

Stiamo andando verso un sistema che concede i pieni poteri. Il collega Amidei dice, giustamente - e tutti i sottofirmatari riconoscono - che il Governo non risponde neanche ai quesiti che i singoli parlamentari, di maggioranza o di opposizione, gli sottopongono. Con l'approvazione dell'Italicum abbiamo messo

terzi dalle scelte del prossimo *leader* di partito e, corrispondentemente, di Governo. La riforma istituzionale limita, demolisce e sminuisce il potere degli enti locali e delle regioni. Mai più ci saranno materie di competenza concorrente, che verranno tutte riavocate e ricentralizzate.

giorni. E ricordo che la tempistica è importante, perché a volte il tempo fa venir meno anche l'esigenza di avere una risposta. È come per la giustizia. Una giustizia che non arriva in tempo è una non giustizia.

conclusione, noi vogliamo dire che il biasimo, a questo punto, non sta tanto nel fatto che non si rispettino i tempi per le risposte. Il fatto è che non si rispetta assolutamente il Parlamento, e ciò significa che non si sta rispettando la Costituzione. È un Governo che deve chiudere

Signor Presidente, oltre a compiacermi del fatto che finalmente in Assemblea si parli di questo tema,

Da un lato, corrispondono alla necessità dei senatori di utilizzare questo strumento come accesso agli atti e come sollecitazione per il Governo. Non dimentichiamoci, infatti, che l'accesso agli atti ha una sua disciplina specifica

È una sollecitazione al Governo non solo per sapere a che punto si è arrivati, ma anche per ricordare ai vari Ministeri di competenza che alcuni territori attendono la realizzazione di atti, magari già predisposti dal Governo stesso. L'altro aspetto, sempre di valore, è

ispettivo è uno strumento d'interazione tra potere legislativo e potere esecutivo e mi permetto di dire che lo è non solo per l'opposizione, ma per tutti

perché l'atto di sindacato ispettivo restituisce in modo migliore il collegamento tra chi dovrebbe fare le leggi e chi le dovrebbe far eseguire o trovare il modo di eseguirle, e poi dovrebbe esserci

certa su questo tema, che riguarda il meccanismo della politica. O vogliamo eliminare completamente l'esistenza di un potere legislativo a fronte di un potere esecutivo, oppure dobbiamo curare quelli che possono sembrare dei fastidiosi inciampi nel collegamento tra i due

sull'utilità di questo strumento e sul grosso rischio che corriamo tutti nell'utilizzarlo in modo indiscriminato. Il problema vero - problema

*(Misto)*. Presidente, le chiedo di rivolgere l'appello al Presidente del Senato di convocare la Giunta per il Regolamento perché ci sia una disciplina diversa. Non è possibile che il ministro Giannini vada al *question time* alla Camera e non venga mai qui al Senato. Non è possibile. Evidentemente qualcosa non funziona

anche in relazione alle rappresentanze territoriali. Vorrei dire alla collega Mussini che la funzione del sindacato ispettivo è in capo a ogni singolo parlamentare, e non si distingue in base a dove è seduto nell'emiciclo quel parlamentare. È un fatto in sé.

qualche intervento, da azioni meramente oppositive dall'utile sollecitazione a fare di più e meglio, che viene a tutti noi e, nella fattispecie, al Governo, che vorrei raccogliere affinché la giornata odierna possa avere qualche elemento di positività ulteriore. Già con la lettera prima e poi con l'interrogazione del senatore Manconi e di altri parlamentari la questione di una maggiore incisività del sindacato ispettivo e, soprattutto, di una maggiore celerità delle risposte era stata posta alla nostra attenzione. Al riguardo ci siamo attivati con doverosa responsabilità nei confronti del Parlamento anche a seguito di ulteriori sollecitazioni. Nel maggio scorso è stata inviata una lettera dal nostro

Nel dicembre scorso vi è stato l'incontro con i responsabili, promosso sempre dal Ministero dei rapporti con il Parlamento, degli uffici legislativi dei vari Ministeri per sollecitare una maggiore celerità.

a parziale confutazione di alcune considerazioni che ho sentito qui svolgere. Il *trend* di risposta agli atti parlamentari dall'inizio di questa legislatura è passato dal 28,6 per

nella legislatura precedente, con il quarto Governo Berlusconi, gli atti presentati sono stati 16.488 e quelli conclusi 6.456;

Ciò che mi pare i dati evidenzino - e mi piacerebbe che, con verità, se ne prendesse atto - è il forte innalzamento degli atti di sindacato ispettivo.

atti che trattano tematiche sensibili per la cittadinanza, questioni di carattere territoriale. Vorrei che comunque si capisse che è complicato dare celere risposta a questo tipo di atti,

nel costruire le risposte che vengono date ai parlamentari. Questo è il tema della complessità, che ha a che fare non con la volontà, ma con una condizione reale.

una maggiore collaborazione. E mi permetto di chiedere che anche gli atti conoscitivi che voi attivate tengano conto di questa reale condizione.

Ovviamente, come Governo non mi posso permettere di intromettermi nell'organizzazione dei lavori. Quello che posso dirvi è che, qualora l'organizzazione cambiasse, siamo assolutamente disponibili a corrispondere alle maggiori e puntuali necessità poste dai colleghi con le mozioni. Per quanto riguarda le mozioni in oggetto, a parte i dati numerici, che ora sono mutati, e e a parte gli impegni o le richieste a cui ho già in qualche modo risposto con questo mio intervento, vorrei dire senatori, se i presentatori sono d'accordo, accoglierei tutte le premesse; suggerirei una modifica nell'ultimo capoverso delle premesse, nel senso di espungere dal testo «è inaudita e inaccettabile, perché», lasciando «Pertanto, la situazione esposta, di fatto, priva i parlamentari»; chiederei di espungere le considerazioni e accoglierei gli impegni. Pertanto, accoglierei integralmente le premesse e gli impegni

Senatore Lucidi, senza arrivare a disturbare il Regolamento, è sufficiente che la Conferenza dei Capigruppo calendarizzi

Signor Presidente, la senatrice Mussini ha ben esposto le questioni, anche di profilo costituzionale,

una seduta, ci sia comunque un problema di convocazione della Giunta per il Regolamento. D'altra parte, le riforme costituzionali sono finite, quindi di che cosa si ha paura? Si può tranquillamente convocare la Giunta per il Regolamento

alle interrogazioni e alle interpellanze, ovvero a tutti gli atti di sindacato ispettivo che abbiamo presentato noi, così come altri Gruppi, altrimenti anche quella di oggi è un'altra giornata che rischia di essere assolutamente persa. Ci attendiamo, quindi, che dalla prossima settimana comincino finalmente ad arrivare le risposte attese.

ed è un'interpellanza del deputato Ferdinando Palluel, dal titolo «L'avvicinarsi delle truppe francesi alla Savoia», scritta peraltro non in italiano, ma in francese. Ebbe risposta il giorno stesso da parte del ministro degli esteri del Regno di Sardegna Pareto, a cui si aggiunsero anche le precisazioni del ministro di grazia e giustizia Sclopis e del ministro dei lavori pubblici Des Ambrois. Da allora le cose sono molto cambiate, come dicevo inizialmente, e i tempi delle risposte si sono prolungati al punto che, per esempio, una mia interrogazione indirizzata il primo anno di legislatura al MISE, esattamente il 5 novembre 2013, sul caso dell'azienda CIL di Livorno, ha avuto risposta nel 2015, ma sopratutto quando non serviva più, perché nel frattempo i lavoratori avevano perso l'impiego. È naturale che se le risposte sono così tardive perdono in gran parte la loro utilità. Nell'arco di due anni molte cose vengono risolte, nel bene o nel male, e l'intervento tardivo del Ministero fornisce informazioni che spesso sono già state da tempo divulgate dalla stampa. A tal proposito, avevo anche depositato un atto di sindacato ispettivo con procedimento abbreviato, sottoscritto da tutto il Gruppo Movimento 5 Stelle, nel quale si chiedeva che il Governo desse risposta agli atti ispettivi presentati, e che ovviamente non è stato preso in carico. Tuttavia, il vero problema che rischia di compromettere definitivamente il delicato rapporto e il dialogo che dovrebbe esserci tra Governo, Ministro e Parlamento, sono le mancate risposte, il silenzio, l'indifferenza. La reiterata mancanza di risposte impedisce e rende impossibile questo dialogo tra membri dell'Esecutivo e parlamentari, e costituisce un ostacolo al funzionamento pieno della nostra democrazia. Come è stato più volte evidenziato nel dibattito parlamentare e in dottrina, alla base del potere di porre interrogazioni e interpellanze vi è un'istanza democratica di cui il Parlamento è il naturale portatore, dato che il nostro ordinamento si configura, appunto, come una democrazia parlamentare. Il potere di porre quesiti riconosciuto ai parlamentari risponde ad un'esigenza democratica e rappresenta una funzione di controllo sull'operato del Governo, riconosciuta fin dalle origini della storia della Costituzione italiana. Nella Costituzione si ravvisa un implicito riconoscimento del potere dei parlamentari di chiedere informazioni al Governo. Nello specifico, l'articolo 64, comma quarto, stabilisce infatti che i membri del Governo hanno diritto e, se richiesto, l'obbligo di assistere alle sedute parlamentari. Questa norma presuppone l'assoluta necessità di un dialogo politico tra i membri del Governo e i parlamentari e ne garantisce la realizzazione, assicurando la partecipazione alle Assemblee parlamentari anche ai membri del Governo. I ritardi e le mancate risposte hanno condotto tutti noi ad avvalerci dello strumento del sindacato ispettivo non per porre quesiti, ma allo scopo di sollecitare risposte ad interrogazioni che non hanno ottenuto risposta: siamo quindi al paradosso. Come si diceva anche prima, sono scandalose le percentuali: 17,9 per cento di risposte alle interpellanze, 29,7 per cento per le interrogazioni a risposta orale, 19,9 per cento per le interrogazioni a risposta scritta. L'Ufficio di Presidenza del Senato, più volte sollecitato affinché tale situazione fosse risolta non è riuscito, come è evidente ad oggi, a porvi rimedio. Molte di queste interrogazioni riguardano semplicemente l'accesso a documenti tenuti in archivio dalle amministrazioni centrali dello Stato. Cioè a volte si richiede solo un documento, un *file* che potrebbe essere inviato semplicemente via *mail*. Ma evidentemente, e sicuramente non nell'interesse dei cittadini e della trasparenza, qualcosa deve rimanere a ingiallire nei cassetti dei Ministeri. Ricordo che più Ministeri si sono rifiutati di fornire informazioni e documenti non sottoposti a particolari vincoli di segretezza, che sarebbero dovuti essere di facile ed immediato accesso non solo per i parlamentari, ma per tutti i cittadini. In molti casi si tratta di documenti che in altri Paesi europei si trovano facendo una semplice ricerca in rete. È da anni che il Ministero della funzione pubblica, almeno a parole, sta portando avanti il progetto di trasparenza della pubblica amministrazione e dei documenti che sono custoditi in archivi di amministrazioni pubbliche. Sarebbe auspicabile avere presto anche in Italia un modello di accesso agli atti della pubblica amministrazione paragonabile alla Svezia o al Regno Unito. Ma forse, per arrivare a ciò, avremmo anche bisogno di un Governo che non aspiri a metodi e modelli autoritari. È evidente che in attesa di una riforma radicale del nostro sistema di accesso agli atti pubblici, i Ministeri potrebbero nel frattempo, agevolare il tutto semplificando i regolamenti interni. Questo semplice intervento garantirebbe immediatamente una diminuzione degli atti di sindacato ispettivo presentati. Resta aperto il problema dell'efficacia delle interrogazioni e interpellanze presentate. Il Governo dovrebbe intervenire affinché siano razionalizzate le strutture e gli uffici che si occupano di rispondere agli atti di sindacato ispettivo. È sconcertante verificare che oltre l'80 per cento di interrogazioni e di interpellanze, orali o scritte, non ottiene alcuna risposta. Gli atti di sindacato ispettivo quale strumento di indirizzo, controllo ed informazione, esistono anche in altri ordinamenti europei, tuttavia risulta che tale arretrato non si riscontra né nel Parlamento del Regno Unito, né presso il Parlamento della Repubblica federale tedesca, né presso il Parlamento della Repubblica francese, Paesi che, per dimensione e complessità istituzionale, sono comparabili all'Italia. In questi Paesi, infatti, i Governi sono riusciti ad affrontare e gestire in modo efficace e razionale tale funzione, perché si sono avvalsi di prassi e strumenti idonei. chiede al Governo di risolvere questa situazione e di non costringerci ad intervenire nuovamente su questo argomento. Personalmente ho presentato circa una sessantina tra interrogazioni e atti ispettivi a risposta scritta e solo due volte ho avuto il piacere di avere risposta. Peccato che le risposte, appunto, le avevo lette mesi prima sui giornali! Non è una questione legata ad un Gruppo politico, si tratta di rispettare le istituzioni democratiche e il dialogo che tra esse deve avvenire. Ricordo che molti interventi di fine seduta dedicati a questo argomento sono stati pronunciati non dai membri dell'opposizione, ma da senatori provenienti dalle file della maggioranza, detto ancora più chiaramente per i cittadini italiani che ci stanno ascoltando, il Governo si rifiuta di rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze degli stessi parlamentari della propria maggioranza. Il Governo, con i suoi Ministeri, dispone di molti uffici. Sarebbe il caso che i funzionari e i dirigenti della Presidenza del Consiglio mostrassero adeguata cura e rispetto per il ruolo che tutti noi ricopriamo.

con le modifiche suggerite dal Governo. Lo riteniamo indispensabile per continuare a svolgere il nostro ruolo, cioè essere la voce dei cittadini. Vedere anche un solo voto contrario sarebbe l'ennesimo campanello di allarme e sarebbe inconcepibile. Un giorno mi è stato regalato un libro da una persona carissima, che si intitola «Lo Stato siamo noi», e per «noi» s'intende tutti i cittadini, il popolo, non un Governo o un soggetto che decide per tutti. Pertanto, invito tutti i colleghi ad unirsi alla nostra richiesta, in nome della democrazia. *(Applausi Signor Presidente, ringrazio il senatore Amidei per avere avuto l'idea di presentare questa mozione, perché lui, a differenza di molti di noi, me compreso, si era abituato a una situazione in cui il Governo ogni tanto risponde. Tutti coloro che sono stati in un Consiglio regionale, provinciale o comunale, sanno che i governi locali, pur avendo indubbiamente molti meno mezzi e meno funzionari che lavorano su queste cose, rispondono. Recentemente ho avuto modo di verificare quanto è stato citato dalla collega: negli altri Paesi i Governi rispondono. I Governi, indipendentemente da quali siano, devono rispondere alle domande, e non farlo una volta ogni tanto, specialmente a quelle che fanno comodo. Le sollecitazioni che consentono di fare un po' di colore alla fine di ogni seduta, nella mia esperienza non servono, purtroppo. Ho sollecitato forse quattro o cinque volte una stessa interrogazione, ma non ho mai avuto risposta,

di rispetto non per il Parlamento, ma per i cittadini. Ci sono alcune cose che dovrebbero essere valutabili attraverso il diritto di accesso. Allora è inutile che ci si presentino delle

cosa. Questa è la situazione che abbiamo avuto fino ad oggi. Apprendo con soddisfazione il fatto che il Governo abbia accettato la parte sostanziale della nostra mozione. Lo prendiamo fermamente in parola, anche i senatori della maggioranza, che immagino voteranno a favore, visto che il Governo ha espresso parere favorevole. L'impegno lo prende anche davanti a voi,

Non a partire da chissà quando, ma a partire dalla settimana prossima, bisogna passare a questa nuova fase, in cui - guarda un po' - alle interrogazioni, come avviene in tutti i Consigli comunali, in tutti i Consigli regionali e in tutti i Parlamenti d'Europa, si risponde.